Signor Presidente, la scorsa settimana, abbiamo approvato la risoluzione relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria.

effetti anche rispetto all'efficacia degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo. Sorge un primo quesito: a quale risoluzione risponderà il Governo, a quella approvata dalla Camera oppure a quella approvata dal Senato?

questi aspetti sia necessario un chiarimento all'interno della Giunta del Regolamento, anche in previsione proprio della Nota di aggiornamento che dovrà essere presentata a settembre. Ritengo che non sia senza significato evitare una contrapposizione tra le due Camere. lei ha assolutamente ragione. È già capitato che non vi sia stata coincidenza nella decisione. Ritengo opportuna una riunione approfondita della Giunta del Regolamento. Per il momento, vediamo come il Governo troverà l'equilibrio

mandandoci in vacanza a metà luglio e ad agosto, anziché continuare a farci lavorare nel periodo meno adatto, senza che nessuno ce lo ordini,

per avere un cenno di assenso o meno a questa che mi sembra una proposta seria, calettata sull'andamento delle temperature, di evitare di vederci trascinare stancamente, con questo caldo terribile, in un periodo in cui sarebbe meglio essere in ferie.

e cioè che il testo della riforma della previdenza dei senatori sarebbe stato distribuito ai senatori prima di essere approvato nel competente Consiglio di Presidenza. A noi è risultato, come le avrà detto il Vice presidente con funzioni di Presidente che era in Aula martedì scorso, che lunedì scorso è stato ufficialmente presentato (ci diceva l'allora presidente Calderoli) consegnandone una copia un'ora prima della riunione, e approvato il testo di riforma della previdenza. Tutti sappiamo che è materia del Consiglio e non è materia dell'Aula, ci siamo permessi di chiedere, con sovrana umiltà, di averne copia prima e non l'abbiamo avuta, ora che è diventato testo ufficiale e che tutti i senatori rispondono al Paese

è stato distribuito ai Gruppi, comunque immediatamente verrà distribuito a tutti i senatori che lo vorranno. Presidente, io mi permetto di sollecitare la sua attenzione in relazione al diritto del Senato ad esprimere il proprio parere in relazione ad un complesso di decreti legislativi che sono stati varati dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso, in attuazione di deleghe contenute nella legge comunitaria

straordinariamente rilevanti, cito tra questi in modo particolare il decreto legislativo che disciplina, recependo appunto la direttiva europea, la materia della lotta al riciclaggio, che introduce disposizioni che limitano fortemente la libertà e la riservatezza delle transazioni anche più minute. Ricordo anche un altro decreto legislativo che amplia le possibilità d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio da parte di cittadini extracomunitari. Ora, il periodo estivo normalmente è computato ai fini del decorso dei termini che sono concessi al Parlamento per poter esprimere il proprio parere (in questo caso si tratta di quaranta la pregherei non solo di interpretare il Regolamento nel senso quanto più favorevole ad un adeguato spazio per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ma d'intervenire anche presso il Governo affinché, in termini politici, si possa determinare uno spazio ancora più congruo. Devo segnalare, con amarezza, che il Governo ha atteso l'ultimo momento utile per l'esercizio di queste deleghe, in qualche modo costringendo anche i tempi dell'esame parlamentare entro limiti oggettivamente molto ridotti. Ma, come ho detto, rimetto alla sua sensibilità la tutela delle prerogative parlamentari a questo riguardo.

e definito il calendario di massima della ripresa dopo la pausa estiva. Oggi pomeriggio, dopo il voto sul parere della 1a Commissione permanente sui presupposti di costituzionalità relativi al decreto-legge in materia finanziaria, sarà tolta la seduta per consentire alla 5a Commissione permanente di proseguire, e possibilmente concludere, l'esame di merito del provvedimento entro l'inizio della seduta antimeridiana di domani, convocata alle ore 9,30. Da quel momento, dopo la relazione e il voto delle questioni incidentali, avrà inizio la discussione generale sul decreto-legge, per la quale sono state ripartite otto ore. La Conferenza dei Capigruppo sarà poi nuovamente convocata, nella giornata di domani, per organizzare il seguito della trattazione e la conclusione del provvedimento. Per quanto riguarda gli altri argomenti da inserire nel calendario di questa settimana, si è al momento convenuto - con decisione che verrà sottoposta ad ulteriore verifica in sede di Conferenza dei Capigruppo - di porre all'ordine del giorno, dopo il voto finale del decreto-legge in materia finanziaria, il disegno di legge recante delega sugli enti di ricerca (già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), per il cui voto finale è richiesta la presenza del numero legale. Sarà inoltre previsto lo svolgimento della sola relazione del disegno di legge collegato sui servizi pubblici locali.

Dopo la pausa estiva, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di mercoledì 12 settembre per la discussione di mozioni sollecitate dai Gruppi. Le Commissioni potranno convocarsi da lunedì 10 settembre, salvo che particolari esigenze dei rispettivi calendari dei lavori non ne richiedano una convocazione anticipata. finestra"). L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,

ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.

ci pone davanti ad un sistema di produzione delle norme giuridiche complesso, perché è composto da due elementi, entrambi necessari: da un lato, il decreto-legge; dall'altro, la legge di conversione. Come dicevo, entrambi necessari, perché il decreto-legge decade senza la legge di conversione, e la legge di conversione non può esistere senza il decreto-legge. La questione nasce su questa domanda: come interagiscono questi due elementi? In particolare, i vizi dell'uno si trasmettono o no all'altro?

la legge di conversione abbia un'efficacia sanante o no nei confronti del decreto-legge. È stata anche presente nella giurisprudenza della Corte, fin dalla prima sentenza che affermò in principio la sindacabilità

sanabilità-non sanabilità - la Corte interviene con la sentenza n. 171 del 2007, stabilendo con chiarezza la non sanabilità. La legge di conversione non sana il vizio della mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza ma, al contrario, questo vizio diventa un vizio in *procedendo* della legge di conversione. Dice la Corte (mi consenta la Presidenza di dare una lettura perché questo comunque contribuirà anche al dibattito in Commissione sul tema): sul tema): «Affermare che la legge di conversione sani in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze parlamentari del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Si

non possono essere valutate sotto il profilo della legittimità costituzionale autonomamente da quelle del decreto stesso». la norma costituzionale, che attribuisce al Governo la responsabilità dell'emanazione del decreto, condiziona nel contempo l'attività del Parlamento in sede di conversione, in modo particolare rispetto all'ordinaria attività legislativa. Da questo, signor Presidente, credo sia corretto dedurre conseguenze in ordine alla necessità di una maggiore attenzione quanto all'omogeneità del decreto-legge: la sentenza n. 171 del 2007 dichiara appunto l'incostituzionalità per l'estraneità della norma presa in considerazione rispetto al contesto. E si richiede maggiore attenzione anche in relazione alla emendabilità, cioè alla possibilità di introdurre nel testo del decreto o anche nell'articolo unico della legge di conversione elementi normativi che siano fuori contesto. Questo è il quadro nel quale si sta svolgendo in Commissione la riflessione. Sui presupposti, in particolare, la Corte costituzionale per la verità non è particolarmente stringente. Dice - leggo un altro passaggio la disposizione costituzionale ha un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può esser dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani, anche atti e provvedimenti dei pubblici poteri), in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi. Voglio sottolineare questo passaggio, signor Presidente, perché mi consente oggi di sostenere in Aula che sussistano i presupposti di necessità ed urgenza, anche per l'articolo 16 che, secondo alcuni colleghi invece presenta dubbi. Mentre - ribadisco - ci vorrà maggiore attenzione da parte sia del Governo nell'adottare il decreto, sia della Presidenza delle Commissioni e dell'Assemblea, nel valutare l'ammissibilità di emendamenti, alla luce di quello che la Corte dice.

A me capita spesso di non condividerle, e per la verità non considero questa Corte una vetta insuperabile del sapere giuridico. Bisogna però fermarsi di fronte ad una sua sentenza. È vero che questo Parlamento è sovrano: ma lo è nel senso che può cambiare la Costituzione o anche ridefinire i poteri della Corte. Essendo la Costituzione quella che è ed essendo i poteri della Corte quelli che sono, nell'attuale assetto costituzionale e normativo, la Costituzione è quel che la Corte decide che sia. Vorrei che questo risultasse chiaro nei resoconti

conclusivamente e pur nell'ambito di una riflessione che dovrà continuare, la conferma della decisione della 1a Commissione favorevole alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto‑legge in esame. *(Applausi dal

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, signor Ministro, io credo che questa discussione cada in un momento estremamente significativo anche se i colleghi rendono difficile non tanto l'essere ascoltati quanto il ragionamento, perché con questo brusìo è difficile ragionare. PRESIDENTE. Colleghi, per favore, ha ragione il senatore Pastore. Il rumore

e fa il paio con la sentenza della Corte che inibì la reiterazione dei decreti-legge. Ricordo ai colleghi quello che accadeva fino a dieci anni fa o poco meno; si reiteravano i decreti-legge, il secondo decreto-legge riprendeva il testo approvato da uno dei rami del Parlamento trasformandolo in norma cogente e così avveniva per due, tre, quattro, fino anche a otto volte. La Corte, a un certo punto, ha detto: basta; per la natura ed il valore della decretazione d'urgenza, per il significato dell'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo questa vicenda deve finire, sapere al legislatore e a tutti gli organi costituzionali che partecipavano e partecipano del processo legislativo del processo legislativo che sarebbe intervenuta, con declaratoria di illegittimità costituzionale, in caso di reiterazione dei decreti-legge. la sentenza di due mesi fa è ancora più drastica rispetto agli effetti di quella sulla reiterazione dei decreti-legge, perché la Corte costituzionale - come ricordava il collega Villone - ha affermato che, ancorché il proprio sindacato sui presupposti di urgenza

signor Presidente, onorevoli colleghi, questa non è una conseguenza di poco conto, non è un'esercitazione giuridica, ma è una conseguenza che impone a tutti gli organi preposti all'esercizio della funzione legislativa (a partire

che la legge di conversione può aver ritenuto sussistenti, stimando che l'intervento del legislatore primario (cioè la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica), in qualche modo, sani questo difetto

però, lei, come Presidente di quest'Aula, e i Presidenti delle Commissioni (innanzitutto, la Commissione affari costituzionali, poi le Commissioni di merito) a svolgere un'attenta riflessione su questa su questa sentenza della Corte. In che misura questa sentenza della Corte può ricadere sul provvedimento in esame? Noi abbiamo chiesto il passaggio in Aula, ritenendo che già nel testo originario mancassero i presupposti di urgenza: mi limito a citare l'articolo 16, in materia di tasse e diritti marittimi, che interviene sul testo di un regolamento,

e politica che ho cercato brevemente di indicare e che nasce da un abuso verificatosi di decretazione d'urgenza, lo stesso che si è determinato per la reiterazione dei decreti‑legge: li abbiamo visti crescere

oltre che di quello della Camera, che richiamano procedure specialissime, proprio perché - ed è questa la premessa e la conseguenza della sentenza della Corte la funzione legislativa appartiene pienamente al Parlamento e il suo esercizio da parte del Governo ha natura eccezionale e quindi deve essere ristretto e limitato negli ambiti della Costituzione,

il messaggio di rinvio alle Camere di un decreto‑legge, approvato nella precedente legislatura, da parte del presidente Ciampi, che richiamò espressamente i contenuti della legge n. 400 del 1988 e che invitò le Camere stesse,

moderò senz'altro la tendenza ad abusare della decretazione d'urgenza. Oggi, questa sentenza della Corte, per quanto controversa, pone un punto fermo credo che chi ha la responsabilità di Governo e ha la maggioranza in quest'Aula e alla Camera debba farsi carico di trovare i sistemi corretti per realizzare quegli obiettivi di Governo che magari questi decreti‑legge, impropriamente ingrassati di norme che non potevano contenere, cercavano di realizzare, attraverso strade diverse da quelle della decretazione d'urgenza. Di questo noi dell'opposizione siamo pienamente consapevoli; non ci tireremo

sono interventi e richiami che devono illuminare e dirigere la funzione di tutte le forze politiche che ai princìpi costituzionali devono attenersi.

sulla sussistenza dei presupposti di urgenza e necessità del decreto‑legge recante disposizione urgenti in maniera finanziaria.

dico questo perché - lo ricordava il collega Pastore nel brusìo generale, come sto facendo anch'io, ma spero che qualcosa alle orecchie dei colleghi possa arrivare, perlomeno per la conoscenza di aspetti delicati che riguardano i rapporti tra Parlamento e Governo e Governo - nel testo del decreto-legge c'è un articolo che, ai sensi della disciplina ordinamentale di livello costituzionale e di livello non costituzionale (quindi, normale ed ordinario),

a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi secondo principi di semplificazione. Praticamente, ci troviamo di fronte a una norma che non può essere contenuta nel decreto-legge

la copertura politica della legge di conversione da parte del Parlamento non fa superare il vizio stesso; anzi, il vizio di legittimità per mancanza dei presupposti si riversa sull'intera legge,

quelle necessarie convergenze, affinché il sistema delle fonti normative del diritto - che è alla base della democrazia del nostro Paese e del nostro sistema politico - possa individuare una soluzione tale, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, che ripristini il valore originario

Spero che l'Aula vorrà fare una riflessione, non tanto per l'approvazione di questo provvedimento, ma per ricercare in futuro soluzioni che siano più rispettose del disegno costituzionale.

anche in queste circostanze, e a sproposito, l'opposizione si è espressa sollevando eccezioni di insussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, che, viceversa, va assolutamente convertito. Esprimo il mio dissenso per quanto ribadito dalle forze politiche opposte e puntualizzo la natura meramente ostruzionistica dell'istanza, che si annovera tra numerose interferenze proposte ad ostacolo del buon lavoro portato avanti finora. L'illustrazione delle ragioni di necessità del provvedimento si coglie semplicemente nella logica in cui vanno attuate queste norme e nel vantaggio indiscusso che ne deriverebbe per gran parte delle categorie delle categorie sociali: occorre cioè dare immediata collocazione alle risorse derivanti dal gettito fiscale, rivelatosi consistentemente superiore alle previsioni. In ogni caso, è facilmente percepibile la finalità del provvedimento, tesa alla tutela concreta degli interessi di una larga fascia sociale e, in special modo, a sostegno dei più deboli. Del resto, puntando alla conversione del decreto-legge n. 81, si realizzerebbe ampiamente il duplice obiettivo di risanare i conti pubblici e fortificare le politiche di sviluppo ed equità sociale. Questo è quanto si è promesso, quanto ci si aspetta dalla manovra, quello che daremo agli elettori. È un segnale forte, in risposta alle attese di molti contribuenti ad oggi molto scontenti, ma che potranno cominciare a percepire i frutti dei sacrifici profusi. Detto ciò, mi pare urgente incrementare le pensioni basse, necessario sostenere le imprese, equo tagliare il cuneo fiscale, opportuno aver dato ascolto agli addetti ai lavori di concerto con le associazioni di categoria per ricucire atavici strappi. Per questi motivi, l'Udeur ritiene oltremodo urgente e necessario procedere nell'*iter* di conversione del decreto-legge. Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, la Lega Nord ritiene il provvedimento

gli interventi annunciati siano eterogenei sia sotto il profilo dei contenuti, sia per quanto concerne l'ambito delle amministrazioni e dei settori considerati:

Il preambolo del decreto-legge afferma, infatti, la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza con riguardo all'esigenza di interventi nei settori più vari,

eterogenei, come la garanzia della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario e il sostegno a vari specifici settori dell'economia. È evidente che tali norme potevano essere inserite

delle risorse a disposizione della struttura commissariale ai fini della conclusione dello stato emergenziale, fornite dal Governo durante la discussione del decreto-legge n. 61 del 2007 in materia.

effetti immediati che tali non possono essere considerati e che fanno cadere i princìpi di costituzionalità limitati perché prevedono una funzione esclusivamente organizzatoria e procedimentale, che rimandano a successivi provvedimenti per le modalità attuative. l'articolo 4 prevede un decreto del Ministro dell'economia che fissi criteri e modalità per i rimborsi previsti (quindi, anche qui non si intravedono i requisiti di necessità ed urgenza); l'articolo 5, in materia pensionistica, prevede un decreto del Ministro del lavoro che determini incrementi, nonché modalità e termini di corresponsione; il comma 7 dell'articolo 6 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio per la determinazione

che anche dagli Uffici viene considerato quantomeno anomalo. Pertanto, rimandiamo a due considerazioni: in primo luogo, la legge di contabilità, all'articolo 11-*ter,* richiede giustamente una variazione normativa *ad hoc* a garanzia della solidità dei mezzi di copertura che non possono consistere in semplici previsioni di maggiori entrate, entrate, e pensiamo che tale norma attuativa dell'articolo 81 della Costituzione debba essere in posizione rafforzata rispetto alla legge finanziaria, per la quale

stabilita per la prima volta nella storia del Senato della Repubblica. Affidiamo, cioè, alla previsione di un DPEF modificato dal Senato,

Qui non c'è più il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione! Tra l'altro, viene previsto come copertura un miglioramento del risparmio pubblico per gli anni 2008 e 2009 senza andare a valutare gli andamenti aggregati, che dovrebbero, come minimo, essere organizzati affinché l'incremento

che la decretazione d'urgenza è una facoltà di normazione primaria che la Costituzione, all'articolo 77, riserva al Governo. È altrettanto consapevole che tale facoltà può essere esercitata quando il Parlamento non è in grado di adempiere utilmente alla sua funzione percorrendo l'ordinario *iter* legislativo. È a tutti noto che il requisito e il presupposto per l'esercizio di tale funzione legislativa del Governo sono la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. che non sia più noto ad una parte di quest'Aula che la necessità non è da confondere con l'opportunità politica e che l'urgenza non è da confondere con la speditezza. Sembra, infatti, che una parte dell'Assemblea abbia confuso questi sinonimi. Vi è da dire che il collega Villone e successivamente il collega Pastore hanno saputo sviluppare - non mi trattengo su questo aspetto - i rapporti tra il decreto-legge e la legge di conversione, alla luce dell'ultima sentenza n. 171, che ha messo un punto fermo sulla questione che per anni ha in varia misura investito la Corte costituzionale.

che si configura anche come conclusione del suo esame, aggiunge un ulteriore elemento peggiorativo alla volontà di esproprio del Parlamento nella sua specifica funzione legislativa. L'impotenza cui è ridotta quest'Assemblea democratica è inoltre dimostrata da altri profili di costituzionalità sulla mancanza dei presupposti di urgenza e necessità. Il primo, più sintomatico, è la disomogeneità di materia. Sembra una minifinanziaria con il compito di incidere sulle poste di bilancio, soprattutto sul lato della spesa, che si qualifica così come una manovra finanziaria senza però la necessità di un intervento sui saldi di finanza pubblica. Tale aspetto è enfatizzato dalle rilevanti modifiche intervenute intervenute in Commissione bilancio alla Camera. Sono stati modificati i contenuti del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Presidente della Repubblica. È stato qui ricordato come quella promulgazione avrebbe dovuto tenere conto dei presupposti di carattere costituzionale di cui oggi stiamo discutendo, ma di cui purtroppo ne rileviamo l'assenza. Questo ulteriore aspetto di esame e di controllo da parte del Presidente della Repubblica è stato oggetto di critica dal centro-sinistra quando era all'opposizione. Più volte i colleghi Villone, Salvi ed altri si sono soffermati su tale aspetto, anche se oggi sembra ne abbiano dimenticato la fondatezza e risultano piuttosto silenziosi: forse hanno cambiato idea oppure si vergognano di questa prassi e tacciono. Un ulteriore elemento di incertezza costituzionale sull'urgenza è rilevabile alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

senza che sia stato ancora approvato il disegno di legge di assestamento del bilancio. Può essere urgente e necessario un decreto-legge che non ha copertura finanziaria? Un principio elementare di contabilità stabilisce che possono essere autorizzate spese se vi sono altrettante entrate a copertura delle stesse.

le maggiori entrate di 7 miliardi e 403 milioni di euro del famoso tesoretto, mentre già se ne autorizza la spesa, stante l'efficacia della normativa riguardante il decreto-legge sul tesoretto in discussione. Finora il tesoretto è una risultanza di cassa, ma non è mai stato riconosciuto come competenza, ossia come misura giuridica di autorizzazione di spesa. come si fa a compiere questo salto logico nel nostro ordinamento. Questa è la domanda che dovrebbero porsi, oltre alle argomentazioni che sono state

che esula dai presupposti di cui stiamo discutendo ma che mi preme sottolineare: esso è rappresentato proprio dalla violazione dell'articolo 117 della Costituzione con riferimento al comma 6 dell'articolo 15 del provvedimento in esame. Si tratta della costituzione del fondo per l'accesso al credito dei giovani. La Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha espresso il proprio il proprio giudizio di illegittimità costituzionale delle varie norme riguardanti i fondi speciali, inserite a varie titolo nelle leggi finanziarie, su materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle Regioni. Qui si seguita pervicacemente ad ignorare un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale; non solo, ma nel caso specifico si ignora la sentenza n. 137 del 2007, riferita al comma 336 dell'articolo 1 della finanziaria 2006 (quella del centro-destra), che aveva ritenuto incostituzionale l'istituzione di un fondo di accesso al credito per i giovani. solo della violazione dei princìpi di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 81, che qui si rileva ai fini dell'applicabilità dell'articolo 77 della Costituzione, ma anche della palese violazione degli articoli 81 e 117 della

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, desidero preliminarmente ringraziare i colleghi Pastore, Saporito, Polledri e Ciccanti per aver posto in Aula la questione di necessità ed urgenza, pressoché all'indomani della sentenza della Corte costituzionale che rivede i criteri all'interno dei quali il Parlamento è chiamato a valutare i presupposti medesimi della decretazione d'urgenza del Governo.

merita - a mio avviso - di essere criticata, ma certamente ciascuno di noi è chiamato a rispettarla ed applicarla in ogni suo punto. Ho avuto occasione di leggere i lavori della Costituente, la quale non intese mai sottoporre ad alcun limite il potere legislativo del Parlamento, ma fissò, con chiarezza, il limite al potere legislativo del Governo con l'articolo 77 della Costituzione, tant'è che la decretazione d'urgenza venne introdotta solo ed esclusivamente nei lavori dell'Assemblea costituente in Aula, mentre era stata addirittura negata in Commissione. Un intervento assolutamente esemplare dell'onorevole Codacci Pisanelli spiegò, in maniera puntuale, che l'azione legislativa del Parlamento aveva una totale autonomia e non si richiamava al cosiddetto *bill* d'indennità, di regime anglosassone, che aveva invece la potestà di dare copertura legislativa alle responsabilità del Governo che aveva emanato provvedimenti di carattere legislativo; tant'è che nessuna norma, né si può far riferimento alle norme regolamentari del Senato e della Camera, prevede alcuna originalità rispetto al procedimento legislativo ordinario. che le sentenze della Corte costituzionale possono essere criticate, ma devono essere rispettate e applicate, per cui dobbiamo tener fede a questo impegno e verificare, punto per punto, la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza nel provvedimento in esame. debbo dire che i rilievi fatti dal collega Polledri agli articoli 4, 5 e 6, comma 7, riguardano, a mio avviso, più la discussione sui presupposti costituzionali, che potremo svolgere domani, che non su quelli di necessità ed urgenza. Si tratta di misure finanziarie che incidono sull'anno in corso; fissarne la data immediata di entrata in vigore vigore è una condizione che i legislatori della Costituente avrebbero riferito ai cosiddetti decreti catenaccio, per i quali appunto la decretazione d'urgenza, quanto ai presupposti, dovrebbe essere uno strumento normale. Può suscitare qualche perplessità

che l'articolo 16 non è di immediata applicazione, ma fa riferimento ad un regolamento che entrerà in vigore il 30 ottobre 2007. io invito i colleghi intervenuti a leggere con attenzione la norma, così come ho fatto io dopo il loro suggerimento, che mi è stato utilissimo per gli studi di questo fine settimana. L'articolo 16 non autorizza il Governo a emanare un regolamento in materia di tasse marittime, ma proroga un termine fissato in finanziaria, già scaduto tre mesi dopo l'entrata in vigore della finanziaria In questo sta la portata normativa di quella norma e, in realtà, se si va a verificare, il contenuto normativo è specularmente lo stesso rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 989, della legge finanziaria. Quindi, un differimento di termini già scaduti con riferimento ad una norma di riordino tributario non può che essere considerato come supportato da quei requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77, primo comma, della Costituzione. La residua portata normativa è quella di far riferimento all'articolo 17, comma 2, invece che al comma 3 della legge n. 400 del 1988, che - a mio avviso - è la correzione di un refuso normativo, posto che parliamo di delegificazione - avremo modo di parlarne domani - per cui è corretto che sia il Governo e non il Ministro con un regolamento ministeriale a provvedere; altri contenuti normativi, oltre ai criteri aggiuntivi dei quali il Parlamento dovrebbe essere ben lieto che siano stati introdotti, non ve ne sono. Sotto questo profilo, invito i colleghi a riflettere sul fatto che ho preso puntuale nota delle loro osservazioni; li ringrazio per avermi dato occasione di fare un puntuale approfondimento su questo tema e posso dire all'Aula, a nome dell'Ulivo, che sicuramente nel provvedimento in esame sussistono i presupposti di necessità e di urgenza e che pertanto la pregiudiziale da loro presentata va avversata, e il voto non può che essere negativo. *(Applausi